Signor Presidente, oggi è la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Diamo alle persone che soffrono di questa patologia un momento di attenzione in più, un pensiero, una carezza. È un segnale importantissimo, in questa prestigiosa Aula, aprire i lavori parlamentari del 2 aprile parlando di questa tematica. Un'indicazione specifica che il Senato e le altre istituzioni non dimenticano persone troppo spesso, purtroppo, bistrattate nella società civile, proprio a causa dei propri disturbi. Probabilmente non c'è modo migliore di inaugurare questa giornata dedicata all'autismo e ai disturbi dello spettro, ricordando l'approvazione, avvenuta all'unanimità pochi giorni fa in Commissione sanità in sede deliberante, di un disegno di legge dedicato. Il Senato, per mezzo della Commissione sanità e grazie al lavoro proficuo di tutti i suoi membri, ha saputo dare un primo segnale concreto e forte di attenzione a chi soffre di tale patologia e alle loro famiglie. Per questo ora è importante che il percorso della legge abbia un *iter* accelerato alla Camera, in modo da giungere, entro tempi brevi, all'approvazione definitiva. Speriamo, tra un anno esatto, in questa stessa giornata, di poter riferire all'Assemblea dei risultati concreti ottenuti dalla legge sull'autismo, che è un provvedimento quadro. serve infatti ad incentivare l'uguaglianza di trattamento della patologia per bambini, adolescenti e adulti nelle diverse Regioni italiane, secondo *standard* di cura e criteri omogenei ed uguali su tutto il Il prossimo aggiornamento dei LEA, nei quali vengono inseriti la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, è l'altro aspetto fondamentale del disegno di legge, oltre agli obiettivi individuati per le politiche regionali. L'autismo si configura come una disabilità permanente, con una serie di caratteristiche specifiche: accompagna il soggetto nel suo ciclo vitale, si manifesta in forme difformi e variabili e, soprattutto, si caratterizza per un funzionamento mentale atipico, tale da richiedere interventi terapeutici e socio-assistenziali particolarmente dedicati. É importante che una legge dello Stato preveda misure d'intervento che vanno dalla diagnosi precoce, alla cura, all'abilitazione in tutte le fasce d'età, con particolare riguardo alla formazione di un approccio educativo-sanitario che sia, per quanto possibile - ce lo auguriamo di cuore - strutturato, completo e organico. Inclusività dei bambini nella società che li circonda tramite una rete di servizi competenti, possibilità concrete di inserimento lavorativo per gli adulti, sostegno specifico alle famiglie: sono questi gli obiettivi generali per fornire alle persone con autismo un futuro che sia il più normale possibile. Tali obiettivi non si perseguono solamente con una legge, pur necessaria, ma occorre soprattutto adoperarsi e lavorare nella comunità per una maggiore consapevolezza sull'autismo, che è innanzitutto I disturbi dello spettro sono molto frequenti, senza differenza di etnie e condizione sociale. Per tale ragione l'autismo è una condizione che richiede un dispendio di risorse umane ed economiche cospicue. Secondo studi approfonditi, le voci di spesa più importanti sono i servizi di educazione speciale e la perdita di produttività dei genitori quando il figlio è in età infantile e adolescenziale, mentre in età adulta i costi maggiori sono legati alle cure domiciliari o alle residenze assistite e alla perdita di produttività individuale. Per dare un'idea dei costi dell'autismo basta ricordare come nel Regno Unito essi siano maggiori di quelli dell*'ictus* e del cancro messi insieme. L'elevata frequenza del disturbo, la sua cronicità e gli alti costi dell'assistenza ne fanno una vera e propria emergenza sociale e sanitaria, non solo nei Paesi occidentali ma in tutto il mondo, ponendo pressanti questioni di politica sanitaria e di ricerca delle molte cause dei disturbi dello spettro, conosciute soltanto nel 20 per cento Per questo oggi si è deciso di dare rilievo internazionale alla giornata sulla consapevolezza e voglio ricordare a questa Assemblea le molte iniziative territoriali, curate da genitori interessati, dalle istituzioni, dalle associazioni, dai ricercatori e dagli operatori, che ogni giorno, nel proprio piccolo, lottano per donare un futuro possibile a persone che soffrono. Oggi dedichiamo loro, ai loro sforzi quotidiani e a tutte le persone affette da autismo e disturbi dello spettro il nostro primo pensiero e le nostre intenzioni migliori.

Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati, ciascuno in *parte qua* per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio)». La relazione è stata stampata e distribuita. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Altero Matteoli nella sua qualità di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore* e delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*; all'unanimità, con separate votazioni, di proporre all'Assemblea di concedere la predetta autorizzazione a procedere in giudizio anche nei confronti dei coindagati Piergiorgio Baita,

per i fatti mi rimetto alla relazione scritta. Intendo però portare all'attenzione dell'Assemblea alcune precisazioni. La legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989 ha riportato i cosiddetti reati ministeriali nell'alveo del rito penale ordinario, bilanciando il principio di parità di fronte alla giurisdizione con quello della garanzia della funzione di governo. La salvaguardia della funzione di governo è attuata in primo luogo attraverso l'attribuzione dello svolgimento delle indagini preliminari al Tribunale dei Ministri e in secondo luogo attraverso l'autorizzazione a procedere di una delle due Camere secondo due cause di giustificazione *extra ordinem* che la Camera competente è chiamata a valutare. Queste due fattispecie sono atte ad evidenziare motivi di ragion di Stato tali da rendere inopportuna la prosecuzione del procedimento penale e si specificano nella tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero nel perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Quindi, la Giunta da me presieduta ha dovuto accertare la sussistenza o meno di una delle due cause di giustificazione *extra ordinem* appena richiamate. La memoria depositata dal senatore Matteoli (come l'altra depositata da uno dei coindagati) incentra il fulcro delle argomentazioni sulle violazioni procedurali commesse - a giudizio della difesa della procura di Venezia, sulla collaborazione assicurata dal Ministro all'autorità procedente, sulla scelta di avvalersi della polizia tributaria e sul *modus operandi* della polizia tributaria stessa, sulle modalità con le quali è stato svolto l'interrogatorio del dottor Mazzacurati, sulla violazione dei diritti di difesa (tra i quali l'impedimento dell'accesso ad alcuni atti di indagine), sulla incompetenza territoriale del tribunale di Venezia, sulla «fuga di notizie», sulle anomalie della relazione trasmessa al Senato, su profili inerenti ai reati ministeriali oggetto dell'accusa ed, infine, sull'illogicità della contestazione della fattispecie corruttiva. Analoga impostazione difensiva è stata seguita dal senatore Matteoli anche nel corso dell'audizione in Giunta. Nella memoria e nell'audizione, pertanto, non emerge alcun nesso tra l'illecito contestato al senatore Matteoli e l'interesse dello Stato o quello pubblico allo svolgimento della condotta criminosa (nella specie, della condotta corruttiva).

atteso che il Senato può decidere solo sulle richieste di intercettazioni inoltrate dall'autorità giudiziaria, ma non su quelle non inviate. In sede di replica, lo scorso 7 gennaio 2015, in Giunta ho chiarito, in qualità di relatore, che il Senato non ha alcuna possibilità oggettiva di far emergere le predette irregolarità procedurali, nemmeno attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione. Ribadisco quindi come il diniego di autorizzazione a procedere, ai sensi della sopracitata legge costituzionale, motivato dalle lamentate violazioni procedurali, sarebbe illegittimo e configurerebbe un vizio di eccesso di potere per sviamento dalle finalità. Nel corso dell'istruttoria compiuta dalla Giunta, non è emerso, infatti, alcun profilo di interesse pubblico al conseguimento illecito delle somme oggetto del patto corruttivo, almeno secondo la tesi investigativa. Il reato, nelle forme in cui sembra essersi perfezionato, rende difficile l'individuazione delle cause giustificative contemplate dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e sulle quali il senatore Matteoli non ha fornito alcuna spiegazione. Ragionando in termini assoluti, intendo sottolineare un passaggio fondamentale: anche qualora la difesa affermasse la propria estraneità ai fatti (nel senso di non averli commessi o di non essersi gli stessi verificati), il sindacato della Giunta si deve esprimere nel senso della autorizzazione a procedere; mentre la "confessione" del fatto operata da un Ministro ma spiegata in ragione delle fattispecie fattispecie *extra ordinem* deve essere valutata dalla Giunta secondo la sussistenza o meno di una delle cause di giustificazione previste dalla legge costituzionale di riferimento. Un elemento, emerso nel corso del dibattito, attiene alla circostanza che, secondo la prospettazione dell'accusa, il senatore Matteoli aveva stipulato degli atti di transazione tra lo Stato e un'impresa responsabile dell'inquinamento a Porto Marghera, attribuendo poi i relativi finanziamenti al Consorzio Venezia Nuova, in relazione alla bonifica dei siti industriali localizzati in tale area territoriale. Secondo quanto sottolineato nel corso della discussione generale da parte di alcuni senatori intervenuti secondo quanto prospettato dallo stesso interessato nella sua memoria, depositata in Giunta), il senatore Matteoli non avrebbe avuto altre opzioni se non quella di dare attuazione alle decisioni della Presidenza del Consiglio precedentemente in carica. In particolare, l'*ex* Ministro dell'ambiente sostiene, nella memoria, di aver dato attuazione alle precedenti determinazioni della Presidenza del Consiglio e, in particolare, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1999, con cui è stato approvato l'accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera dell'ottobre del 1998. Alla luce di tale ricostruzione, è stata prospettata da alcuni colleghi intervenuti la configurabilità della causa di giustificazione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, ossia il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Tale assunto, però, non è condivisibile, in quanto negli atti trasmessi dalla procura si legge testualmente che «Matteoli Altero riceveva denaro contante direttamente da Mazzacurati e Baita per l'importo di euro 400.000 e di euro 150.000 consegnati per il tramite di Colombelli William Ambrogio e di Buson Nicolò». Il reato, nelle forme in cui sembra essersi perfezionato, non può essere giustificato dall'interesse pubblico governativo, atteso che l'ipotetica necessità di dare legittimamente attuazione ad una decisione del Governo precedentemente in carica non giustificherebbe comunque il senatore Matteoli rispetto alla presunta (sottolineo presunta) ricezione di una somma di denaro per l'esercizio di tale funzione. Nel corso del dibattito, alcuni senatori intervenuti hanno infine sostenuto che l'ipotesi di corruzione, oggetto dell'accusa, non è riconducibile in alcun modo alla fattispecie dei cosiddetti reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione, per cui è stata prospettata la necessità da parte della Giunta di dichiarare la propria incompetenza e deliberare, pertanto, la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria. Tale soluzione coinciderebbe a mio avviso, sotto l'aspetto pratico, con l'autorizzazione a procedere. Sul piano teorico, tuttavia, la tesi della non riconducibilità della fattispecie in questione all'articolo 96 non è stata accolta, in quanto il *pactum* corruttivo nel caso di specie è stato stipulato in relazione all'esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici spettanti al senatore Matteoli, in qualità di Ministro *pro tempore*. Per questi motivi e per i motivi che più dettagliatamente sono esposti nella relazione, la Giunta, come lei ha testé detto all'Assemblea, nella seduta del 7 gennaio 2015, ha assunto le seguenti deliberazioni: accolto, a maggioranza la proposta per l'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore* e delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*; ha accolto invece all'unanimità, con separate votazioni, le proposte per l'Assemblea di concedere la predetta autorizzazione a procedere anche nei confronti dei coindagati Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo

per brevità e per non annoiarvi, non ripercorrerò nel dettaglio la vicenda giudiziaria che mi vede coinvolto. Questa è una sede politica e istituzionale che non è chiamata a giudicare nel merito. Tuttavia, nel momento in cui si chiama in causa non più il semplice cittadino Altero Matteoli, bensì l'*ex* Ministro dell'ambiente e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, credo sia giusto che il Senato abbia piena contezza delle questioni che vengono sottoposte al suo esame, con particolare riferimento a talune anomalie e violazioni costituzionali che sono state riscontrate anche nel corso dell'esame del fascicolo nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Vengo ai fatti: nel maggio dello scorso anno mi venne recapitata una lettera dalla procura di Venezia nella quale si comunicava l'apertura di un fascicolo senza oggetto definito. Dopo non poche difficoltà, i miei legali riuscirono ad ottenere copia degli atti ed appresero che nell'ambito della nota inchiesta sul MOSE di Venezia il principale testimone di accusa, di nome Mazzacurati, presidente del Consorzio Venezia Nuova, aveva dichiarato di avermi personalmente remunerato con denaro e finanziamenti elettorali per i favori a lui fatti nel corso degli anni. Altri testimoni, che non ho mai avuto modo di incontrare né di conoscere, affermavano che i favori da me fatti al consorzio sarebbero consistiti nel trasferimento al magistrato delle acque di Venezia, struttura del Ministero delle infrastrutture, dei fondi che il Ministero dell'ambiente era riuscito ad ottenere dalle imprese ritenute responsabili dell'inquinamento di Porto Marghera. A fronte di queste accuse, ho avuto modo di dimostrare che l'unico finanziamento elettorale ricevuto dal consorzio, pari a 20.000 euro, è stato immediatamente restituito dal mio committente elettorale al mittente. È negli negli atti e ci sono le contabili bancarie. Non è assolutamente smentibile quello che sto dicendo. Ho chiesto di potermi confrontare con il Mazzacurati per conoscere in quale circostanza avrei mai ricevuto dal medesimo del denaro contante. Ho anche fornito all'autorità giudiziaria i miei estratti conto degli ultimi dodici anni e tutte le informazioni riguardanti le mie disponibilità patrimoniali perché, anche sotto questo profilo, non c'è davvero nulla da nascondere. Ho consegnato persino ai magistrati le matrici degli assegni emessi dal 2004 alla fine dell'anno 2014. Ma tutto questo è materia processuale e l'approfondimento in quella sede l'avremo certamente. Non posso invece fare a meno di rilevare che ai miei legali è stato negato il diritto di interrogare il Mazzacurati, sebbene gli stessi si fossero dichiarati disposti a partecipare all'interrogatorio in qualunque momento ed in qualunque luogo. Il Mazzacurati è stato sentito per rogatoria negli Stati Uniti d'America dove si trova a suo dire per gravi problemi di salute e, nel corso di un interrogatorio che definire surreale è un puro eufemismo, ha affermato, contraddicendosi platealmente rispetto a precedenti deposizioni, che mi avrebbe dato soldi in due occasioni.

oppure nella mia abitazione di Lucca. Ma, signori colleghi, io a Lucca non ho mai avuto casa: tutti possono acclarare che io non ho mai avuto a Lucca una casa né di proprietà né in affitto.

con l'espressione: «Ma no, buttate via tutto», riferendosi alle risposte appena rese. È molto importante, onorevoli colleghi, spiegare quale sia stato il comportamento tenuto

correttamente il relatore il Ministero dell'ambiente diede attuazione alle precedenti determinazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri (in particolare, al decreto del 12 febbraio 1999 del Presidente del Consiglio) con le quali era stato approvato l'accordo di programma sulla chimica

il magistrato delle acque e l'autorità portuale di Venezia provvedessero alle preliminari e necessarie opere di conterminazione dei siti e che il magistrato delle acque realizzasse, anticipandone la spesa, gli gli interventi di marginamento dei canali industriali nell'area di Porto Marghera, provvedendo poi - cito testualmente - «a ripetere quanto anticipato presso le aziende che risultassero, in sede giurisdizionale o transattiva responsabili dell'inquinamento». Pertanto, da Ministro dell'ambiente mi sono mosso, com'era mio preciso dovere, esclusivamente per attuare precedenti decisioni del Governo, nella specie, oltretutto, di altro colore politico, conferendo addirittura dei fondi ricavati dalle transazioni ad un Dicastero diverso dal mio. alle valutazioni della Giunta, che qui sono state ricordate solo in parte. Nell'ambito dei lavori della Giunta è emersa la violazione di diverse norme costituzionali e processuali nel corso delle indagini. Di tali circostanze si è discusso con chiarezza in Giunta.

«le rilevanti violazioni di regole procedurali e costituzionali commesse nel caso di specie dalla competente procura», evidenziando che in uno Stato di diritto il mancato rispetto delle leggi non può essere giustificato in nessun caso, nemmeno quindi per il perseguimento di un determinato fine. Il senatore Alicata ha evidenziato che «nel caso di specie sono ravvisabili clamorose violazioni di norme procedurali, anche di matrice costituzionale». ha sottolineato che «nel caso di specie sono state commesse da parte dell'autorità giudiziaria violazioni costituzionali gravissime, rispetto alle quali il Senato non può restare indifferente», «sia con riguardo alle intercettazioni illegittimamente effettuate sia relativamente all'ingiustificato ritardo con il quale sono stati trasmessi gli atti

«la lamentata effettuazione di intercettazioni in violazione dell'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione (di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989)», sottolineando che «qualora la Camera competente ritenesse che l'autorità giudiziaria procedente abbia leso la sfera delle proprie attribuzioni riconosciute dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, potrebbe anche sollevare il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale», ma lamentando al contempo la difficoltà di «effettuare un'adeguata ricognizione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l'attivazione del conflitto nel caso *de quo*». Dagli atti del procedimento si evince, inoltre, che la procura della Repubblica di Venezia non ha tempestivamente trasmesso l'incartamento che mi riguarda al Tribunale dei Ministri, ovvero entro 15 giorni come prevede la legge costituzionale, bensì con ben nove mesi di ritardo durante i quali la polizia giudiziaria non si è astenuta dal proseguire le indagini, contravvenendo ad un esplicito divieto posto dalla stessa legge costituzionale. Altra anomalia: sono state effettuate, in modo del tutto illegittimo, ben 213 intercettazioni telefoniche indirette sulla mia indirette sulla mia utenza telefonica per le quali mai è stata avanzata richiesta di autorizzazione al Senato. Preciso di non avere mai avuto, e non ho tutt'ora nessun timore: usino pure le

Presidente, io le ho fatto pervenire una nota di due autorevoli costituzionalisti che hanno messo in evidenza questo ma non per difendere me stesso, perché Matteoli si difenderà nelle aule giudiziarie, bensì perché lei prenda contezza di questo per tutelare i senatori. Non è possibile che un magistrato possa effettuare delle intercettazioni senza autorizzazione. di non avere alcun timore ed alcuna preoccupazione riguardo ai contenuti di tali intercettazioni che dimostrano, al contrario, la mia assoluta correttezza; ma sta di fatto che esse sono state realizzate e poi utilizzate a fini probatori in modo del tutto illegittimo. A tale proposito, ho ritenuto di sottoporre alla Presidenza del Senato l'autorevole parere di due illustri costituzionalisti, perché al di là del caso specifico del senatore Matteoli, ritengo che su questi temi ci debba essere la dovuta attenzione. Varie sentenze della Corte costituzionale hanno stabilito che possono essere utilizzate, senza autorizzazione, le intercettazioni indirette di un parlamentare solo se esse sono sporadiche e casuali. Non mi pare che 213 intercettazioni si possano considerare sporadiche e casuali.

Infine, è fin troppo evidente l'incompetenza territoriale di Venezia rispetto ad accuse che fanno riferimento ad ipotetici reati commessi a Roma oppure in Toscana, ed anche questo tema - particolarmente serio e delicato - merita di essere conosciuto e considerato. le mie richieste, alla luce di queste circostanze, taluni colleghi mi hanno rappresentato la loro intenzione di presentare ordini del giorno per chiedere il respingimento della proposta della Giunta - ho qui i testi che sono a mio avviso correttissimi per la sussistenza del presupposto del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della mia funzione di Governo. Altri colleghi hanno evidenziato la possibilità che il Senato promuova un conflitto di attribuzione per far valere le proprie prerogative. prerogative. Ringrazio i colleghi per aver manifestato l'attenzione rispetto a queste problematiche, che non attengono solo alla forma, ma anche alla sostanza della vicenda giudiziaria. altresì ringraziarvi, colleghi, per avere accolto il mio invito ad evitare qualsiasi iniziativa che potesse far sorgere delle ombre sul mio operato di cittadino, di parlamentare e di Ministro.

Sin dal sorgere di questa storia surreale incredibile e, allo stesso tempo, sconcertante, ho pensato, superando le forti resistenze dei miei avvocati e degli amici, che la via migliore sarebbe stata quella di non prestare in alcun modo il fianco all'imperante populismo, che spesso negli ultimi tempi è degenerato in autentiche aggressioni mediatico-giudiziarie contro la classe politica del Paese. Io desidero sottopormi comunque al vaglio della giustizia, ai suoi accertamenti che, sono certo, saranno svolti con professionalità e indipendenza di giudizio. Chiedo pertanto, signor Presidente, che l'Assemblea del Senato, come prescrive il Regolamento, dia per accolte le conclusioni cui è pervenuta a maggioranza la Giunta, ossia che autorizzi la magistratura a procedere nei miei confronti. Io mi difenderò con determinazione e forza, perché non ho nulla da temere. È mia precisa volontà, cari colleghi, affrontare a testa alta questa vicenda nella certezza che tutto potrà essere chiarito nelle aule di giustizia con piena soddisfazione del sottoscritto e di chi, in oltre trent'anni di permanenza nell'agone politico, ha creduto nella mia onestà e nella trasparenza dei miei comportamenti nelle varie responsabilità pubbliche che ho avuto ed ho l'onore di ricoprire.

Non troverete mai scritto sui giornali che Altero Matteoli ha patteggiato: non patteggerò mai niente, a nessun costo. Non si patteggia ciò che non si è commesso.

per il ruolo che ha svolto prima di essere senatore - avranno notato che alcuni reati o ipotesi di reato

io non ho nulla da ammettere, per cui non posso patteggiare. Insomma, voglio difendermi nel processo, non dal processo, continuando a godere, se possibile, della stima e della fiducia di coloro che mi conoscono.

giudici di merito e la Corte di cassazione potranno certamente dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata acquisizione dell'apposita autorizzazione se dirette.

Presidente, ho preso atto della richiesta del senatore Matteoli di non presentare ordini del giorno alternativi, perché così ha voluto, nonostante vi fosse una chiarissima indicazione da parte del tribunale dei Ministri che vi era stato uno sviamento di potere non corretto perché perché si era adeguato a quanto stabilito dal presidente D'Alema. Detto questo però, non sono intervenuto per questa ragione, ma perché il Presidente della Giunta delle elezioni